L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Onorevoli colleghi, comunico che l'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulla manovra economica, già prevista per le ore 12, avrà luogo alle ore 13. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 13.

Presidente, Gentile Presidente, onorevoli senatrici e senatori, nel riferire al Parlamento sugli esiti del dialogo con la Commissione europea, desidero in primo luogo esprimere il mio sentito ringraziamento a tutti voi, di maggioranza ma anche di opposizione, per la comprensione mostrata in questi giorni durante i quali l'*iter* di esame del disegno di legge di bilancio ha proceduto con lentezza, scontando un ritardo rispetto ai tempi previsti. I rinvii non sono stati causati - come sapete - da incertezze interne alla maggioranza di Governo. Nei giorni scorsi, si è imposto un rallentamento del vostro esame, così determinando una inevitabile compressione del dibattito in Commissione a causa della complessa interlocuzione che è intercorsa con l'estensione dell'Unione europea, alla quale abbiamo dedicato le nostre più risolute energie e il nostro più intenso impegno. Questa interlocuzione ci ha richiesto inesorabilmente molto tempo come è inevitabile, d'altra parte - in un negoziato caratterizzato da forti connotazioni politiche, seppur dipanate lungo il binario di un serrato confronto tecnico di natura finanziaria e contabile. In queste settimane, durante le quali i canali del dialogo non si sono mai interrotti, abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni, senza mai arretrare - desidero rimarcarlo - rispetto agli obiettivi che, con il voto del 4 marzo, gli italiani hanno ritenuto prioritari nell'azione di Governo. Come è noto, allo scopo di rispondere alle urgenze e ai bisogni avvertiti dai cittadini e dalle imprese, abbiamo realizzato interventi di equità sociale, di inclusione e di sostegno al reddito che, in base a una stima iniziale, hanno determinato, insieme alle altre misure anche di investimento, un *deficit* del 2,4 A fronte della decisione del Governo, la Commissione europea ha espresso le proprie riserve, preannunciando l'avvio, nei confronti dell'Italia, di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. Si profilava così per il nostro Paese una prospettiva che andava evitata. Abbiamo lavorato con la massima determinazione per evitare la procedura di infrazione, dialogando a più riprese con il Presidente e alcuni componenti della Commissione europea in particolare, ma anche con vari Capi di Stato e di Governo di singoli Paesi membri, al fine di illustrare ai nostri interlocutori il più ampio disegno riformatore e di persuaderli sulla opportunità di giungere, nel reciproco interesse, a una soluzione condivisa. Abbiamo pienamente salvaguardato la nostra impostazione della manovra di bilancio.

Proviamo

Non abbiamo ceduto sui contenuti, certi degli effetti virtuosi che nel medio periodo una manovra espansiva potrà determinare sul tessuto economico e sociale e comunque fermi nelle determinazioni...

...fermi nelle determinazioni assunte con il contratto di Governo, cioè rispondere all'esigenza, fortemente avvertita, di invertire le politiche di rigore che negli anni passati hanno aggravato la crisi, determinando una forte compressione dei redditi, una riduzione dei consumi, un generale impoverimento di ampie fasce della popolazione.

Quando il 21 novembre scorso la Commissione ha formalizzato le sue riserve sulla versione rivista... sulla versione rivista del documento programmatico di bilancio presentato dall'Italia, i margini di negoziazione sono risultati subito davvero contenuti ed esegui. È stato allora che, con il sostegno dei Vice Presidenti, dei Ministri, e del Ministro dell'economia in particolare, mi sono assunto l'onere e anche la responsabilità di riannodare i fili del dialogo affinché non fosse compromesso il processo riformatore che il Governo intendeva realizzare già con questa sua prima manovra economica. Ho dunque insistito con il presidente Junker perché si rendesse disponibile a un ulteriore incontro, che si è svolto sabato 24 novembre, nel corso di una cena di lavoro a cui hanno partecipato anche il ministro Tria, il vice presidente della Commissione e responsabile per l'euro e per il dialogo sociale Dombrovskis, e il commissario degli affari economici e monetari Moscovici. In quell'occasione ho presentato l'ampio progetto riformatore del Governo, chiedendo ai miei interlocutori che la manovra economica fosse valutata non solo al filtro dei vari saldi contabili, ma più ampiamente alla luce dell'articolato spettro di interventi - alcuni già realizzati, altri in fase di avanzata elaborazione - tutti tesi a semplificare, migliorandoli, i rapporti tra Stato, cittadini e imprese. In quella sede - come pure in ulteriori incontri avvenuti informalmente a margine del G20 a Buenos Aires ho potuto registrare alcune rigidità di posizioni, ma allo stesso tempo - devo dirlo - anche alcune significative aperture al dialogo. All'esito di queste interlocuzioni, si è reso necessario uno sforzo ulteriore da parte del Governo per verificare la percorribilità di interventi utili a migliorare i saldi finali contenuti nella legge di bilancio, in adesione ai rilievi formulati dalla Commissione. Abbiamo quindi lavorato affinché fosse puntualmente quantificata, con apposite relazioni tecniche, la stima economico-finanziaria delle misure, soprattutto di quelle a carattere sociale e previdenziale, che avevano maggiormente attirato l'attenzione dei nostri interlocutori europei. Queste valutazioni, che hanno richiesto tempo, hanno rivelato che le risorse effettivamente necessarie per la realizzazione dei due principali interventi erano - e sono - inferiori a quelle inizialmente previste. Ciò ha permesso di ridurre il disavanzo dal valore inizialmente stimato del 2,4 per cento ad un valore attestato intorno al 2,04 per cento, senza per questo modificare, né nei contenuti - attenzione!

Desidero ribadirlo: reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno nei tempi che avevamo previsto. Con queste nuove quantificazioni quantificazioni mi sono recato a Bruxelles mercoledì scorso, 12 dicembre, per un nuovo confronto con il presidente Juncker e con i commissari Dombrovskis e Moscovici. In quella sede, come pure nel corso di alcuni colloqui con vari *leader* europei a margine del Consiglio che si è tenuto il 13 e il 14 dicembre scorsi, ho ribadito la necessità che lo sforzo compiuto dal Governo italiano per giungere a un punto di equilibrio e di convergenza non fosse frustrato da un approccio che tenesse in esclusiva considerazione il rigido computo degli scostamenti. All'esito di ulteriori interlocuzioni, fino ai risolutivi colloqui di ieri mattina, che hanno portato ad un significativo avanzamento nella trattativa, ho formalizzato la posizione dell'Italia con una lettera ai vertici della Commissione europea, sottoscritta insieme al ministro Tria, che mi ha affiancato in questa complessa trattativa. Nella lettera, oltre a riferire sulle nuove quantificazioni delle misure di spesa, ho rilevato che le modifiche dovranno necessariamente tenere conto dell'evoluzione del quadro macroeconomico, che evidenzia, ahimè, un conseguente peggioramento, principalmente dovuto al cattivo andamento del commercio internazionale. Il rallentamento del ciclo economico impone adesso un aggiornamento delle previsioni di crescita, con l'indicazione di un PIL programmatico all'uno per cento per l'anno prossimo, con una variazione che si ripercuote

Nell'ambito delle misure adottate per la riduzione dei saldi di bilancio, indicati dalla manovra di finanza pubblica, prevista nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021, al fine di corrispondere alle richieste formulate dalla Commissione europea in sede di esame del documento programmatico di bilancio, in primo luogo, come già ricordato, sono state affinate le misure contenute nel disegno di legge di bilancio, anche al fine di determinare con maggiore precisione l'esatta portata degli interventi predisposti e delle coperture individuate. Grazie a questa attività è stato possibile rivedere l'onere annuo delle misure di cui al fondo per il reddito di cittadinanza e quello per gli interventi pensionistici, mantenendo integro - lo ribadisco - l'impatto concreto di queste due misure. Sono state poi previste misure di contenimento della spesa pensionistica, che si sostanziano nel raffreddamento dello schema di indicizzazione dei trattamenti pensionistici di più cospicuo importo. Inoltre, si interviene sulle cosiddette pensioni d'oro, con una riduzione dei trattamenti più elevati, attraverso la previsione di un contributo di solidarietà temporaneo e progressivo per scaglioni di reddito: una misura di equità sociale, da cui abbiamo ricavato ulteriori risorse. Sono stati quindi quantificati gli effetti dell'utilizzo in via prioritaria da parte delle Regioni delle risorse già stanziate nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la realizzazione degli interventi di mitigazione dei rischi ambientali e idrogeologici. Si introducono, inoltre, misure per favorire la realizzazione del piano straordinario di dismissioni immobiliari. Sul lato delle entrate si prevede la revisione delle clausole di salvaguardia IVA per gli anni 2020-2021, l'istituzione di un'imposta sui servizi digitali gravante sui soggetti che, nell'esercizio di attività di impresa, prestino servizi digitali e che superino determinate soglie di ricavi, l'abrogazione anche del credito d'imposta relativo alle deduzioni forfettarie in materia di IRAP riconosciute in favore di soggetti passivi che impiegano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in alcune Regioni; l'abrogazione del credito d'imposta in favore di soggetti che compiono investimenti in beni strumentali nuovi, l'abrogazione dell'aliquota ridotta IRES in favore degli enti non commerciali, un pacchetto di misure che incrementa il prelievo nel settore dei giochi attraverso l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento e la riduzione delle percentuali minime di *pay-out*. inoltre, dal 1° gennaio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le amministrazioni centrali si prevede un rinvio della presa di servizio degli assunti al 15 novembre 2019, ma limitato alle assunzioni derivanti dal *turnover* ordinario dell'anno precedente. Si è tenuto conto, inoltre, della stima di maggiori entrate contributive per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in relazione alle quote di risorse stanziate per l'attribuzione al reddito di cittadinanza e destinazione all'assunzione di personale destinato a rafforzare le attività dei centri dell'impiego. Sono state, altresì, inserite alcune riduzioni e riprogrammazioni della spesa che non necessitano di modifiche alla sezione 1 del disegno di legge sul bilancio. In particolare, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste misure volte a definanziare le risorse del fondo per favorire lo sviluppo del capitale immateriale, la competitività e la produttività di 75 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per l'anno 2020. Abbiamo, inoltre, programmato una rimodulazione delle disponibilità di cassa del fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale destinato a misure per il superamento degli squilibri socio-economici-territoriali per 800 milioni di euro per l'anno 2019. Tengo a chiarire Tengo a chiarire che questa riprogrammazione coinvolgerà la concreta spendibilità e non pregiudicherà in alcun modo la realizzazione di tutti i progetti già programmati e anche dei nuovi che potranno tranquillamente essere programmati. Su questo punto c'è l'impegno pieno - come sapete - di tutto il Governo e la responsabilità mia personale anche a intervenire in corso di anno per recuperare eventuali risorse suppletive che, casomai, dovessero rivelarsi necessarie. Allo stesso modo, abbiamo programmato una rimodulazione delle risorse finanziarie per 600 milioni di euro per l'anno 2019 prevedendo un incremento, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, di 200 milioni di euro delle risorse destinate alla società Ferrovie dello Stato per la realizzazione di progetti previsti. Abbiamo previsto, infine, una rimodulazione con riduzione di 850 milioni di euro per l'anno 2019 e un incremento progressivo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 di 150 milioni di euro e per l'anno 2025 di 100 milioni di euro della quota nazionale per il finanziamento delle politiche comunitarie. anche per queste due ultime voci vi è il pieno impegno del Governo e ribadisco la mia personale responsabilità affinché tutti gli interventi già programmati siano realizzati, se necessario, anche attraverso interventi di recupero di risorse suppletive. L'ammontare dei saldi, così ridefiniti, è, dunque, pari a 10.254 milioni nel 2019,

ho rappresentato anche l'esigenza di approntare un piano di interventi straordinari per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie (viadotti, ponti, strade, gallerie) e la gestione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico. Per questi interventi il Governo ha chiesto e ottenuto che sia applicata la flessibilità prevista dal Patto di stabilità e crescita, in misura - pensate - corrispondente a quasi lo 0,2 per Questo piano straordinario ci consentirà di tutelare più efficacemente l'incolumità dei cittadini e di mettere in piena sicurezza il territorio della nostra penisola, realizzando una sequela di rapidi interventi secondo un cronoprogramma prestabilito. A tale piano saranno dedicate risorse già appostate in bilancio negli esercizi precedenti, per vari investimenti, e anche parte delle nuove risorse disponibili dalla legge di bilancio in corso di approvazione e dal decreto-legge in materia fiscale collegato alla manovra economica. Nel 2019 si utilizzeranno complessivamente risorse per 2 miliardi e 600 milioni circa. Per gli anni successivi si prevede di spendere, fra risorse già appostate in bilancio e nuove risorse, circa 3,7 miliardi nel 2020 e oltre 4 miliardi e 200 milioni nel 2021, per un totale di 10 miliardi e 500 milioni. Relativamente alla rete viaria e di collegamenti italiana, il crollo del ponte Morandi a Genova ha evidenziato la necessità di intraprendere un programma di manutenzione straordinaria. Nel 2019 saranno dedicati a tal fine 1 miliardo e 100 milioni di euro fra risorse nuove e risorse già appostate in bilancio. L'implementazione effettiva degli interventi sarà oggetto di uno specifico e attento monitoraggio, secondo le stesse modalità previste per la generalità delle opere pubbliche e delle opere in particolar modo cofinanziate dall'Unione europea. Infine, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio, il Governo italiano sottoporrà al Parlamento una norma che dispone l'accantonamento temporaneo di una parte di alcuni specifici stanziamenti, per l'importo complessivo di 2 miliardi. Le somme accantonate saranno rese disponibili nel caso in cui, in corso d'anno, il monitoraggio dell'andamento dei conti evidenzi che esso è coerente con gli obiettivi programmatici. Abbiamo sempre detto che la nostra manovra è rigorosa e conseguentemente rigoroso sarà anche il monitoraggio. Questo, in sintesi, è il quadro compiuto e definito degli interventi che hanno determinato un miglioramento dei saldi finali contenuti nel disegno di legge di bilancio, passando dal 2,4 per cento al 2,04 del rapporto *deficit*-PIL per il prossimo anno,

il loro impatto sul tessuto non solo economico e produttivo, ma, se mi permettete, anche sociale del Paese. Possiamo dire in coscienza di aver realizzato appieno il mandato conferito dai cittadini, dimostrando determinazione nell'esercizio delle prerogative di politica economica che spettano al Governo italiano, di avere perseguito con pieno senso di responsabilità una soluzione condivisa, buona per gli italiani e soddisfacente anche per l'Europa A fronte dello scostamento inizialmente consentito, inidoneo al raggiungimento degli obiettivi programmati, abbiamo varato una manovra economica espansiva che prefigurava uno scostamento di molto superiore. All'esito di una trattativa serrata, condotta con tenacia e determinazione con le istituzioni dell'Unione europea, abbiamo raggiunto un punto di equilibrio sostenibile, attestandoci su uno scostamento che rimarca oggettivamente un valore comunque superiore a quello che la Commissione riteneva idoneo per chiudere la trattativa senza rischiare l'avvio della procedura d'infrazione. La Commissione ha risposto questa mattina trasmettendo, pochi minuti prima delle ore 12 (ed è la ragione della richiesta di rinvio di questa una comunicazione nella quale, prendendo atto delle misure di bilancio che il Governo intende sottoporre al Parlamento, assicura che l'adozione di queste misure permette alla Commissione stessa di non raccomandare l'avvio di una procedura per disavanzo eccessivo.

Ho ritenuto doveroso intervenire in Senato immediatamente dopo l'invio formale della comunicazione e riferire a questo consesso l'informazione appena ricevuta.

L'azione di Governo

L'azione di Governo può adesso proseguire a ritmo pieno, senza gli effetti pregiudizievoli che una procedura d'infrazione avrebbe comportato per l'esercizio delle prerogative di politica economica che legittimamente spettano a un Governo che voglia realizzare un significativo cambiamento nell'ambito della vita politica, economica e sociale del Paese.

Formulo a tutti voi l'augurio di buon lavoro e, vista l'imminenza delle festività, anche gli auguri di buon Natale.

sollevati dal raggiunto accordo con l'Europa, che speriamo sia formalizzato il prima possibile e sentiamo di ringraziarla per la tenacia con cui lei e il ministro Tria avete portato avanti questo delicatissimo La procedura d'infrazione sarebbe stata una mazzata micidiale per la tenuta dei conti pubblici e la fiducia degli investitori e dei risparmiatori. Tuttavia, non possiamo dimenticare

come conseguenza l'aumento dello *spread*, il quale, come ci ricorda l'ABI, ha già avuto effetti sulla vita reale delle persone, con un aumento del tasso medio dei nuovi mutui e del credito per le imprese. Senza il braccio di ferro, non ci sarebbe stato il fatto che un ramo del Parlamento sia stato costretto ad approvare una manovra provvisoria e che il Senato, a dodici giorni della fine dell'anno, non sia ancora stato messo nella possibilità di discutere di discutere il nuovo provvedimento che perverrà nelle prossime ore. Questo tempo sarebbe stato essenziale per costruire una manovra che guardasse con grande convinzione alla crescita e allo sviluppo, una necessità quanto mai impellente, davanti a un orizzonte macroeconomico che non lascia ben sperare. Per noi questo resta il punto più dolente dell'intera manovra. È vero che alla Camera sono state apportate migliorie, ma, come ha calcolato la CGIA di Mestre, è una manovra che nel complesso sottrae sottrae risorse al sistema produttivo. La Commissione bilancio, della quale faccio parte anch'io, avrà solo quarantotto ore per lavorare sul testo. Ci comporteremo con responsabilità, la stessa che abbiamo avuto in questi giorni, quando abbiamo atteso in vano che la Commissione potesse svolgere i propri lavori. Nelle poche ore a disposizione, ci impegneremo per consolidare quelle parti della manovra e del testo che guardano alla crescita e allo sviluppo. stessa responsabilità che lei, signor presidente Conte, ha mostrato nella trattativa con l'Europa e che ci aspettiamo - e che continueremo ad aspettare - da parte di tutti gli esponenti del suo Esecutivo, ringraziando

Signor Presidente, non è mai troppo tardi per agire con responsabilità, soprattutto quando in ballo vi siano i conti e la credibilità di un Paese intero.

a tutelare gli interessi del nostro Paese e non condividiamo la politiche a volte burocratiche e sbagliate di austerità della Commissione europea. Abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità in questi giorni, a fronte del fatto che non era e non è stato possibile discutere di nulla in relazione alla legge più importante per il nostro Paese. senso di responsabilità, non possiamo non sottolineare come siamo arrivati qua per un insieme di gravissimi errori che il Governo ha scaricato sul Paese sulla credibilità dell'Italia, mettendo il Parlamento nelle condizioni di votare alla Camera una legge che non c'era e di non discutere qui al Senato. Sinceramente, signor capisco il suo imbarazzo a fronte del fatto che il Ministro dell'interno fa le politiche degli esteri, a fronte di dichiarazioni che lei deve inseguire. Capisco il suo imbarazzo, tuttavia, dall'avvocato del popolo ci saremmo aspettati un soprassalto, un esercizio di verità. E invece no: continua la stucchevole retorica del Governo del cambiamento, degli impegni elettorali e della campagna elettorale senza soluzione di continuità, tutto sulla pelle degli italiani. Presidente, se vi siete sbagliati a fare i conti sui costi di quota 100 e reddito di cittadinanza,

Oppure, se non è così (e non è così) allora, Presidente, quando direte la verità? Quando direte che non siete in grado di corrispondere alla propaganda?

tutto quello che è stato detto. Io vi consiglierei, anche per un fatto di propaganda, di dire di più: non 4 miliardi e mezzo per il reddito di cittadinanza ma 6,7.

disegno di legge di bilancio con grande serietà e grande impegno, senza far perdere un'ora perché noi l'esercizio provvisorio non lo vogliamo: prima di tutto l'Italia. Tuttavia, voi avete perso una grande occasione perché quello che avete fatto da ultimo si poteva fare qualche settimana fa. Si poteva accogliere il ragionamento di ridurre il *deficit*, di cambiare il denominatore. Tutti gli istituti del mondo vi hanno detto che

per l'ambiente, per la messa in sicurezza. Su questi temi, Presidente, avremmo fatto una battaglia con lei per metterli fuori dal Patto di stabilità e avremmo insieme, come Italia, cercato di affermare i valori del Paese. Non ce l'avete consentito, pensando di giocare al gioco delle tre carte, ma gli italiani, Presidente, lo capiranno e purtroppo dovremo a quel punto verificare cosa significa l'accantonamento di 2 miliardi

evitato una procedura d'infrazione sul debito che avrebbe significato consegnare l'Italia nella prigionia per sette anni della Troika europea.

L'assenza pesa molto più delle false parole dette e delle false promesse annunciate, ripetute dei falsi numeri circolati per mesi in quest'Assemblea, a Palazzo Chigi e anche nei documenti ufficiali. Le assenze pesano. pesano. Abbiamo evitato la prigionia, ma siamo in libertà vigilata perché ora siamo monitorati dalle istituzioni europee per gli impegni che la sottoscritta in questi giorni per una manovra FI-BP)*. Una manovra inesistente, una manovrina da quattro soldi; non c'è nulla in questa manovra. Abbiamo già pagato un prezzo altissimo in termini di *spread;* 5 miliardi in più il prossimo anno il costo per lo Stato, in termini di risparmio, di mutuo e di credito alle imprese. Un prezzo altissimo per nulla. Mi spieghi, Presidente, come può ancora definire questa manovra espansiva se lei stesso prevede che il prossimo anno la crescita del PIL sarà forse dell'uno per cento. A quanto ammonterà la crescita

può esserci una manovra espansiva senza crescita? Per i provvedimenti di cui parlate (per quel provvedimento che ha fatto esultare il Vice *Premier,* qui assente, che aveva addirittura annunciato la fine della povertà in Italia,

ricordo che nei documenti del Movimento 5 Stelle il reddito cittadinanza costava 17 miliardi. L'avete detto voi per anni ai cittadini, avete preso i voti su questo punto, parlando di 17 miliardi per il reddito cittadinanza. A quanto sono ridotti?

Con i soldi del REI, 2 più 4, si arriva a 6. Non sono 17 miliardi, ma 6, compresi i due che già venivano dati per sopperire alla povertà; una mancia elettorale pari

Avete copiato il provvedimento nella speranza di gabbare gli elettori come ha fatto Renzi. Questo non è il Governo del cambiamento,

di tassare le pensioni del ceto medio, cioè di chi ha lavorato, prodotto e pagato i contributi, quando si parla di rimodulare

Lì abbiamo calcolato 5 miliardi in più di tasse per le imprese; con quelle che qui dobbiamo dedurre, da quanto già annunciato, andiamo ben oltre. Questa è una manovra che tassa chi produce, che tassa chi ha prodotto, scippando della propria pensione chi ha pagato i contributi, che tassa l'Italia che lavora per fare cosa? Appena un decimo delle risorse è destinato agli investimenti. Sapete quanto avete destinato alla ricerca, al futuro? 64 milioni di euro. Sapete quanto avete destinato all'università? 54 milioni di euro. È una manovra finta, inesistente, fatta sulle spalle del futuro degli italiani, solo per dispensare promesse elettorali. Ciò che conta per voi è che sia in vigore per aprile. Perché per aprile? Perché inizia la campagna elettorale. E che cosa leggiamo sui giornali? Che i due Vice *Premier* sono convinti, non dai numeri, ma dai sondaggi: guardate solo ai sondaggi e alla campagna elettorale, svendendo il Paese. Signor Primo Ministro, non avete abolito la povertà, non avete abolito la corruzione, non avete abolito la mafia: avete abolito la verità. Fate un decreto in cui abolite la verità. D'altra parte questa manovra, nella sua inesistenza, per quel poco che fa, tassando chi produce e cercando di distribuire qualcosa a chi non lavora - e lo dico misurando le parole la prima manovra comunista della storia d'Italia. e, come tale, finirà per abolire la verità. Ma la verità non può essere abolita: si ritorce contro tutti e contro l'Italia e la recessione che è alle porte è tutt'altro che espansione, significa decrescita triste e infelice. Dobbiamo cambiare: rispetto alla Caporetto che si è profilata, bisogna il prima possibile fare una linea del Piave. Dobbiamo farlo per la necessità del Paese, dobbiamo farlo per il futuro del Paese. Signor Presidente, ogni falsità è una maschera e, per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre a distinguerla dal volto. Per la prima volta, signor Presidente del Consiglio, per quanto lei si sforzi, lei qui è nudo, senza la maschera. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lei è qui, peraltro, perché noi l'abbiamo obbligata a venire.

allora il nastro di questa pellicola, che - ahimè - non vincerà alcun premio. Era il 28 settembre quando il suo vice presidente Luigi Di Maio si affacciava dal balcone di Palazzo Chigi, con la faccia stravolta, per festeggiare l'intesa raggiunta sulla manovra al 2,4 per cento del PIL. Di Maio la definì la «manovra del popolo», che per la prima volta nella storia di questo Paese avrebbe cancellato la povertà

con tasse diminuite al 15 per cento per più di un milione di lavoratori e diritto alla pensione per almeno 400.000 persone. Le parole d'ordine erano tutte contro l'Europa. Di Maio, forte della sua arroganza politica, disse addirittura: «Il 2,4 non si tocca, altrimenti faremo cadere il Governo». Lei, presidente Conte, ricorda che cosa è accaduto dal giorno dopo? È successo che i mercati sono impazziti, che lo *spread* è schizzato alle stelle superando costantemente quota 300 punti base. Lo ricorda, Presidente? Mi permetta quindi una domanda, forse ingenua: chi paga i danni che avete prodotto in quei giorni di follia allo stato puro? Perché avete ingaggiato un braccio di ferro con l'Europa intestardendovi su dei valori che non potevate permettervi e sapevate di non potervi permettere? L'avete voluta definire «manovra del popolo»: preciso. Mai più precisi, signor Presidente: è proprio la manovra del popolo, perché mai come oggi è proprio il popolo a pagare. Ha il coraggio di dire agli italiani che, nel bel mezzo di questa vostra irresponsabile recita, ci sono 50.000 posti di lavoro in meno in questo Paese? Che stiamo pagando un miliardo e mezzo in più di interessi sul debito e che sono aumentati di conseguenza i mutui per le imprese e le famiglie? Ha il coraggio di dire che la produzione industriale è calata e che l'Italia tende alla decrescita? Ecco, mentre accadeva tutto ciò in questi mesi, voi siete passati dalla guerra all'Europa al cappello in mano. È successa una cosa incredibile: dai *Diktat* fortissimi e feroci contro l'Europa, siete finiti a farvi scrivere la manovra, virgole comprese, da quelli che chiamavate i tecnocrati di Bruxelles. Avete avviato una prima lettura alla Camera completamente falsa, un testo ancorato ancora al 2,4 per cento che, dal giorno successivo all'approvazione a Montecitorio, è diventato carta straccia. Poi siete venuti a balbettare al Senato. Bruxelles non vi aveva ancora corretto il compitino e intanto i giorni passavano e voi non sapevate cosa dire di fronte ad un ritardo che aveva e che ha dell'incredibile. È letteralmente la prima volta che la legge più importante dello Stato ha una natura completamente extraparlamentare e viene scritta riga per riga

Sa, questo luogo si chiama «Senato della Repubblica», presidente Conte, e questo luogo aspetta ancora le risposte che fino ad ora lei non ha dato. Lei ci deve dire chi paga i miliardi dati in fumo per la vostra follia. Ci deve dire quali tagli avete operato per rispettare gli ordini della Commissione europea: 10 miliardi in meno di quanto avevate propagandato nei giorni scorsi. A breve avremo forse l'onore, finalmente, di poter leggere la vostra manovra (più che vostra, quella di Junker). Ne parleremo nelle prossime ore, però nulla potrà più cambiare il giudizio del Partito Democratico su questa pagina nerissima del Governo: un giudizio drastico, perché il suo, presidente Conte, lo dico con rispetto, senza maschera è il volto di un pugile affaticato che non è finito al tappeto semplicemente perché ha lasciato il *ring*; il problema è che ha lasciato l'Italia fuori dal *ring*, a scappare da quel *ring*. *(Applausi dal Nella vita tutto è perdonabile, ma lei è il Presidente del Consiglio, e al Presidente del Consiglio del nostro Paese non potremo mai perdonare di avere in soli sei mesi compromesso l'immagine di un Paese stimato da tutto il mondo per la sua umanità

ringraziamo innanzitutto il Presidente del Consiglio e il Governo per questa informativa. Ci viene da dire che finalmente ci siamo trovati davanti a un negoziato con l'Europa e anche questo è un segno importante di cambiamento dei tempi, visto che eravamo abituati, in passato, a seguire con troppa remissività le decisioni della Commissione europea. è stato intenso, è durato anche per un lungo periodo ed è la testimonianza che l'Italia ha giocato la sua partita senza sottomettersi.

Cosa ci dà la misura del fatto che non ci siamo sottomessi? La circostanza che i commissari europei oggi, durante la conferenza stampa, abbiano detto che è stata evitata la procedura di infrazione ma la soluzione adottata non è proprio quella ideale per l'Europa. Questa è la testimonianza

più care al nostro Esecutivo (ovviamente mi riferisco a quota 100 e al reddito di cittadinanza). Grazie per aver ridato dignità - ed è questo che il popolo oggi sente, dopo aver dopo aver seguito tutte queste trattative - ad un Paese abituato a subire le scelte dell'Unione europea e che invece oggi viene considerato con maggiore rispetto. Ricordiamo che siamo partiti dall'1,6

se è vero il detto *melius abundare* *quam* *deficere*, quando si fanno le manovre, bisogna farle con intelligenza.

Chi ha pagato i danni delle politiche di *austerity* che hanno eliminato la classe media del nostro Paese?

senza rinunciare alle nostre priorità: già e, sapete, è anche un bel segnale all'Europa ed ai mercati che tutte le balle che avete raccontato sul fatto che vogliamo uscire dall'Europa non sono vere. Noi non vogliamo uscire dall'Europa; vogliamo cambiare le regole comuni

oggi bisognerà riconoscere - perché questo è ciò che il popolo italiano farà, e lo dovrete riconoscere anche voi - le sue doti di ottimo mediatore e negoziatore, per aver giocato un ruolo decisivo per il nostro Paese.

difficoltà di Governo e di rapporti internazionali. Avremmo potuto facilmente mettere in scena manovre ostruzionistiche; avremmo voluto occupare quest'Aula del Senato per protestare contro l'evidente spoliazione del Parlamento e delle sue funzioni. Il Parlamento, presidente Conte, è il popolo, quel popolo che tanto - spesso - a torto viene invocato in quest'Aula dai partiti che sostengono il suo Governo. In nome della sovranità nazionale - pensi un po' - avremmo voluto occupare quest'Aula, perché è evidente che la manovra che l'Assemblea dovrà frettolosamente approvare a scatola chiusa, sotto forma di maxiemendamento - persino con un voto di fiducia non è la manovra che avreste voluto fare. È la manovra che vi è stata dettata negli uffici e nelle stanze della Commissione europea. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Non lo abbiamo fatto perché siamo responsabili; non l'abbiamo fatto perché l'Italia rischiava - e temo tuttora rischi - una procedura di infrazione; il che vuol dire consegnare le chiavi della politica economica del Paese per i prossimi anni a signori che vivono a Bruxelles, piuttosto che a Francoforte. Non lo abbiamo fatto - forse avremmo dovuto farlo - per amor di Patria, lo stesso amor di Patria che oggi ci obbliga a a porle delle domande, presidente Conte. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Sapendo che abbiamo alle spalle tre trimestri di crescita negativa, e sapendo che il quarto trimestre ragionevolmente non sarà di segno diverso rispetto ai tre che l'hanno preceduto,

ed è questo che forse avrebbe colpito e impressionato la Commissione europea. Invece no. Invece avete fatto una manovra puramente clientelare, volta unicamente a massimizzare i risultati elettorali dei due partiti che sostengono questo innaturale Governo in vista delle prossime elezioni europee. Questa, presidente Conte, è una colpa che non può essere taciuta in questa Aula; una colpa che temo risuonerà nelle strade e nelle piazze del Paese nei prossimi mesi, probabilmente nei prossimi anni. Perché poi, sapendo - per esperienza storica e per intelligenza politica - che picchiare i pugni non serve e che isolarsi nel contesto europeo per difendere l'interesse nazionale non porta i frutti sperati? Lo sappiamo, lo sapete, avreste dovuto capirlo. Tsipras in Grecia e il grande Hollande in Francia non hanno fatto gli interessi del loro popolo; hanno danneggiato i loro popoli. allora quando si scriveva il DEF i suoi due Vice *premier* - oggi stranamente assenti - ancora teorizzavano di sfondare il 3 per cento di *deficit*? Perché nelle interviste continuavano a dichiarare guerra all'Europa? Perché non avete scritto una manovra di sviluppo? Perché avete continuato con questo atteggiamento di aggressione rispetto alla Commissione europea, che tanto è sembrato essere strumentale, come per avere un nemico oggettivo, un argomento da campagna elettorale? Perché avete sistematicamente ignorato i mercati finanziari per poi finire per accucciarvi

ammesso che «Nord» si possa ancora dire - e il MoVimento 5 Stelle. Ora manca il collante, mancano l'identità e il futuro. Io la penso come il ministro Paolo Savona che non credo sia un pericoloso vassallo dell'Europa, un servo dei cosiddetti poteri forti. Paolo Savona ha cercato all'inizio, evidentemente senza riuscirci, di violare i parametri europei e di rompere i *Diktat* europei ma in ragione di una manovra che creasse effettivamente sviluppo; non essendoci riuscito, è arrivato alla conclusione che, non potendo cambiare la manovra, l'unica cosa sarà cambiare il Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Noi di Forza Italia attendiamo ardentemente che questo cambiamento, l'unico cambiamento di cui il Paese ha bisogno, si consumi.

Signor Presidente, Signor Presidente del Consiglio, colleghi, io ho invece la sensazione che per vedere cambiare questo Governo dovremo aspettare almeno altri quattro anni e mezzo, perché anche in questa circostanza il Governo ne è uscito rafforzato portando gli interessi dei cittadini sui tavoli europei.

Avremo modo nelle prossime ore di entrare nei dettagli della manovra, ma voglio sottolineare una questione perché le recenti cronache dei nostri vicini a quanto capitato in Francia - ci dimostrano che quando le istanze dei cittadini, le loro preoccupazioni e le loro frustrazioni non vengono intercettate dalla politica si tramutano poi in tumulti di piazza, in difficoltà e città

esiste infatti un saldo contabile e finanziario che non tenga conto del saldo sociale; non esiste l'equilibrio finanziario, senza un equilibrio sociale che sia possibile. allora che questa manovra dimostri invece che si possono tenere assieme le necessità di bilancio e le necessità economiche di un Paese. La limitazione

con la quota 100, ma ci sono poi tante altre cose, nei tanti emendamenti che anche le forze di maggioranza hanno proposto all'interno del disegno complessivo della legge. C'è la questione dell'abbattimento delle tabelle INAIL, che dà un grandissimo segnale di abbattimento del costo del lavoro; c'è ovviamente la *flat tax*, che consentirà a 900.000 partite IVA di avere un'imposizione fiscale inferiore; c'è un miliardo e mezzo per i truffati dalle banche. Ci sono tante cose e tanti segnali, segnali, che abbiamo messo all'interno di questa manovra proprio per rispondere alle istanze dei cittadini che hanno voluto questo Governo e che hanno grande fiducia in questo Esecutivo e nel suo operato, signor Presidente. Una volta finita questa seduta, dopo aver sentito le sue parole, ci riuniremo in Commissione bilancio e inizieremo l'analisi del dettaglio della manovra di bilancio. Però lo facciamo con una consapevolezza in più: la consapevolezza che quando lei in quest'Aula ha detto di essere l'avvocato dei cittadini le sue non erano soltanto parole. Lei ha dimostrato, in queste trattative, che aveva come primo obiettivo quello di essere a difesa dei diritti dei nostri cittadini che hanno scelto questo Governo. Grazie, signor Presidente.

quando iniziava la fase più feroce del regime nazifascista, i rappresentanti della resistenza valdostana e piemontese delle valli alpine (Emilio Chanoux, Ernesto Page, Osvaldo Coïsson, Gustavo Malan delle valli valdesi piemontesi, Giorgio Peyronel e Mario Rollier) si ritrovarono clandestinamente a Chivasso, in Provincia di Torino, con l'intento di ragionare sul futuro assetto dell'Italia e dell'Europa. Il loro lavoro produsse un importantissimo documento, la Dichiarazione dei rappresentanti delle valli alpine (o Dichiarazione o Carta di Chivasso), che preconizzava la caduta dei regimi nazifascisti in Europa e proponeva la creazione di un sistema politico federale e repubblicano su base regionale e cantonale, nell'insieme di una nuova Europa, anch'essa una federazione di genti, costruita sul rispetto e sulla valorizzazione di tutte le culture e di tutte le minoranze. Grazie, nell'Aula di questo Senato della Repubblica è quello di rimarcare la necessità di riprendere i valori fondanti di libertà e rispetto, i valori della Resistenza, che sono poi i princìpi della nostra Costituzione repubblicana, per ridare vigore a una nuova azione politica, soprattutto in previsione dell'appuntamento elettorale europeo e in un momento storico nel quale i principi e i valori sui quali si dovrebbe basare l'azione politica stanno evaporando. Quindi, una nuova spinta a valorizzare le esperienze e le culture di tutti i territori del nostro Continente, come elemento indispensabile per una nuova e più robusta azione politica, che si orienti verso un vero e proprio federalismo dei popoli. Condizione indispensabile per garantire dignità, giustizia, rispetto e democrazia a tutte le espressioni umane dei territori del nostro Paese e della nostra Europa. Che la Carta di Chivasso, quindi, contribuisca a scuotere le nostre coscienze, in un momento storico di grandi incertezze, di violenza e di iniquità verso un mondo di pace e di giustizia.

Signor Presidente, colleghi senatori, il 12 novembre 2018 sul Bollettino ufficiale della Regione Campania appariva un provvedimento sconcertante: la chiusura la chiusura dei punti nascita dei presidi ospedalieri di Polla, di Sapri e di Vallo della Lucania; vale a dire lo smembramento di questi presidi ospedalieri che insistono in aree perlopiù interne della provincia di Salerno, aree corrose da un fenomeno di spopolamento che sta determinando un'irreversibile destrutturazione demografica di questi territori.

è stata tanto incisiva quanto diffusa ed ha preso, per fortuna, un canale legalitario, non sconfinando in atti di violenza ed illegalità, proprio perché il Senato è stato vicino a queste popolazioni nella persona del presidente della Commissione igiene e sanità, professor Pierpaolo Sileri.

in visita ispettiva, ha verificato la casistica clinica, che non offriva nessun rischio per le partorienti, per i nascituri e per i neonati, ha interagito con i direttori sanitari, ha dialogato con il personale medico e paramedico, si è reso conto delle condizioni orografiche di quei territori, dell'isolamento e dei tempi di percorrenza che esponevano le partorienti e i nascituri - essi sì - a grave rischio della salute e ha concluso la visita con una relazione consegnata al Ministro della salute. il governatore De Luca, messo alle strette, è stato costretto a rimangiarsi i provvedimenti e si è salvata la continuità operativa dei presidi ospedalieri. La cosa che più sconvolge, signor Presidente, è che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 199 del 15 novembre 2018, censura la Regione Campania, nella persona del Governatore commissario, per non avere centrato l'obiettivo del risanamento finanziario: un pieno fallimento!